L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Governo sulla situazione nei Territori palestinesi». Nel dibattito che seguirà alle comunicazioni ciascun Gruppo avrà a disposizione dieci minuti. Al Gruppo Misto sono attribuiti quindici minuti complessivi.

A poche ore dall'annuncio della conclusione dell'operazione «Nubi d'autunno», lanciata all'inizio della scorsa settimana dall'esercito israeliano per contrastare il lancio di razzi Qassam sulle città vicine al confine, un bombardamento d'artiglieria nella zona di Beit Hanun ha colpito, nelle prime ore di ieri mattina, un edificio civile di proprietà della stessa famiglia, uccidendo nel sonno almeno 19 persone, di cui otto bambini e quattro donne, e ferendone 50, 14 delle quali in maniera grave. La dinamica del massacro - causato da un proiettile di artiglieria - non è ancora del tutto chiara, ma sull'evento il ministro della difesa Peretz ha ordinato l'apertura immediata di un'inchiesta. Nel contempo, è stata annunciata l'interruzione di tutte le azioni dell'artiglieria israeliana nella Striscia di Gaza. Il ministro D'Alema ha immediatamente definito «inaccettabile» l'accaduto, ribadendo come «la violenza indiscriminata serva soltanto a seminare odio» e ha auspicato la fine delle operazioni militari e una forte iniziativa internazionale per la ripresa del dialogo. Questa dichiarazione del Ministro è l'ultima di una serie di posizioni e di iniziative prese per raffreddare le tensioni e rilanciare il processo di pace. Il ministro per il commercio estero e per le politiche europee Emma Bonino, in visita a Tel Aviv, ha colto l'occasione per esprimere direttamente al ministro degli esteri israeliano Tzipi Livni la costernazione e la preoccupazione dell'Italia per l'accaduto. Il primo ministro israeliano Olmert ha espresso il suo rammarico per le vittime e ha offerto all'Autorità palestinese assistenza umanitaria urgente e cure mediche per i feriti. Il ministro degli esteri israeliano Tzipi Livni, in una dichiarazione alla stampa, si è rammaricata per le vittime innocenti, ma ha ribadito la consueta posizione del Governo israeliano, secondo la quale le vittime civili dipendono dalla tattica delle milizie palestinesi di farsi scudo, così dice, della popolazione per portare a termine le loro operazioni. Il *premier* palestinese Haniyeh ha condannato duramente il massacro, ha sospeso i negoziati con il presidente Abbas per la formazione di un Governo di unità nazionale ed ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Analoga condanna è venuta dal presidente Abbas, che ha pure invocato l'intervento del Consiglio di sicurezza. L'annunciata interruzione dei negoziati tra Hamas e Fatah per la formazione di un Governo di unità nazionale è forse la conseguenza politica più grave dell'incidente. La creazione di una nuova compagine governativa che incorpori nel suo programma i princìpi del Quartetto (riconoscimento di Israele, rinuncia al terrorismo e rispetto degli accordi sottoscritti dall'OLP) rappresenta infatti il prerequisito per il riavvio dei contatti con Israele. È auspicabile che tale decisione sia frutto solo di una reazione immediata e comprensibile di fronte alla particolare gravità dell'accaduto. La creazione di un Governo di unità nazionale è infatti ancor più necessaria oggi, in un contesto di tensione, nel quale appare fondamentale che tutte le forze politiche palestinesi presentino a Israele un interlocutore istituzionale riconoscibile, accettato e responsabile. Il rischio di una degenerazione della situazione è grave, è inutile dirlo. Naturalmente, non si sono fatte attendere le prese di posizione da parte dei *leader* di Hamas. Appelli della sua ala militare hanno invitato «i musulmani del mondo» a «colpire il nemico americano». Altri esponenti del partito, a partire dal *leader* Khaled Meshaal, residente in Siria, hanno lanciato appelli alla vendetta sul territorio di Israele. Nella Knesset diversi deputati dell'opposizione hanno duramente condannato il massacro. In Israele il dibattito politico sulla crisi è vivo e mostra che possono esistere le condizioni affinché maturi un approccio alla crisi meno conflittuale e più realistico. L'Unione Europea ha già espresso la sua inequivocabile condanna per questo massacro. Essa ha, a mio avviso, nuovi spazi di azione e nuove responsabilità. Intendo ora svolgere qualche riflessione politica più generale.

La Presidenza finlandese dell'Unione Europea ha fatto pervenire il discorso che pronuncerà a nome dell'Unione affinché lo vedessimo per tempo e si tratta di un discorso assolutamente condivisibile. Esprimiamo cordoglio, orrore e una riflessione: in Libano abbiamo spento l'incendio. Per questo si deve ringraziare l'impegno degli europei e in particolare dell'Italia, ma se l'incendio non si spegne a Gaza e in Cisgiordania può di nuovo riaccendere le fiamme in Libano; questo è evidente a tutti. Non siamo in Libano per pacificare il fronte est di Israele e per consentire che sul fronte ovest accada quello che sta accadendo. Il Libano è il punto di partenza e non di arrivo; si deve allargare un processo di pace a cerchi concentrici, perché, come sappiamo, tutto si tiene in Medio Oriente. Il primo cerchio concentrico, dopo il Libano, è quello della Palestina. L'ho detto prima: è necessario un Governo di unità nazionale che è stato bloccato dalla strage; in Medio Oriente c'è chi fa dietrologia, sostenendo che la strage aveva esattamente la volontà di bloccarlo. Abbiamo bisogno di un Governo di unità nazionale, del rafforzamento della fiducia reciproca, passo dopo passo, della fine delle azioni israeliane, della fine del lancio di razzi Qassam, rilascio del caporale israeliano catturato, della riapertura stabile dei valichi di Rafah e Karni, dello scongelamento dei proventi doganali dell'Autorità palestinese, attualmente detenuti da Israele. In questo modo, con queste misure di *confidence building*, si può avviare una trattativa per il processo di pace, che ha l'obiettivo di sempre: due popoli, due Stati. Non c'è altra strada. Lo sanno tutti, proprio tutti; prima si fa,

Occorre affrontare il problema del Golan, quello delle fattorie di Shebaa, che in Libano ha un valore simbolico importante, occorre sapere che Teheran è un *key player* della regione perché esercita la sua influenza su Hezbollah ed anche su Hamas e perché la pacificazione dell'Iraq è impossibile senza un minimo di collaborazione da parte di Teheran. Non è vero che c'è tempo. Non c'è tempo. Se nel 2007 non si avvia l'inizio di una svolta positiva, ci sarà una svolta negativa: si aprirà la strada non alla pace, ma ad una guerra ancor più generalizzata. Abbiamo negli Stati Uniti un nuovo interlocutore, che è il Congresso americano. Presidenza e Congresso americani insieme, in modo *bipartisan*, possono premere su tutti, anche su Israele, per avviare un processo di pace che è urgentissimo. L'Europa ha bloccato la tragedia libanese, ma questo non basta, non è che un punto di inizio se non si riesce ad andare avanti sul percorso della pace.

Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, credo che le prime parole non possano che essere di solidarietà per le vittime di questa nuova, tragica vicenda, di preoccupazione vivissima per gli errori che di tanto in tanto si ripetono e che causano disastri come questo, ma anche di allineamento totale sulle posizioni che l'Unione Europea ha assunto ormai da molti anni in relazione alla vicenda mediorientale e che, anche in questo caso, sembra decisa a portare avanti. Il senso di un intervento, in una circostanza come questa, non può non richiamare la globalità della vicenda palestinese con l'obiettivo unico - forse l'ultimo che ci resta - di non abbandonare la speranza in una pace ancora possibile. In questo caso il nemico peggiore è la rassegnazione ad eventi a volte imprevedibili, ma sempre catastrofici, che potrebbero portare quasi ad un'assuefazione al dolore, al sangue e magari all'idea che una crisi come questa non possa trovare sbocco. Ecco perché mi permetto di richiamare questo sentimento di speranza verso una pace possibile, ricordando anni in cui essa appariva non solo possibile, ma addirittura vicina, a portata di mano,

Erano anni di forte carisma sulla scena mediorientale per due grandi protagonisti: Yasser Arafat e Yitzhak Rabin. I primi, forse, ad avere trovato le parole e lo spirito necessari per avviare un dialogo costruttivo. Rabin nel 1992 venne eletto per la seconda volta *leader* del partito laburista e poi Primo ministro. Dopo alcuni incontri segreti ad Oslo con Arafat, il 13 settembre 1993, a Washington (credo che quella fotografia simbolica sia ancora stampata nella mente e nel cuore di tutti noi), i due *leader* firmarono davanti al presidente Clinton quella dichiarazione di principi che valse non soltanto l'avvio di una stagione proficua sul piano del dialogo, ma anche un riconoscimento fortemente simbolico, come l'assegnazione del premio Nobel per la pace ad Arafat, Shimon Peres e lo stesso Rabin. In quel momento la vicenda palestinese sembrava avviata veramente verso un percorso molto promettente. Il *leader* palestinese Arafat cominciò ad incontrare anche riconoscimenti ufficiali, quelli che gli servivano per portare avanti il suo progetto di realizzare uno Stato palestinese; fino ad allora, infatti, si parlava di Organizzazione per la liberazione della Palestina, ma qualcuno timidamente incominciava a parlare di Palestina come Stato. come sappiamo, la storia è impietosa: uno stop improvviso e drammatico arrivò il 4 novembre 1995, quando, durante un raduno di massa a Tel Aviv su un tema significativo "sì alla pace, no alla violenza", un certo Amir, un estremista di destra israeliano, uccise Rabin. Non a caso, sicuramente, al funerale di Rabin accorsero in massa Capi di Stato e di Governo, non solo per una partecipazione al dolore, ma anche per segnalare che quell'evento non aveva soltanto derubato uno Stato del suo *leader*, ma anche un progetto del suo principale protagonista. infatti, fu il primo ad essere indebolito e ad accusare il colpo. Allora egli rivolse, con grande decisione e determinazione, ogni suo sforzo verso l'Unione Europea. Capì subito - fu quella una mossa importante - che dall'Unione Europea, dall'Europa, non solo per una questione di banale vicinanza geografica, potevano arrivare al suo progetto la spinta e la legittimazione, che gli avrebbero consentito di portarlo fino in fondo. Il Parlamento europeo istituì una delegazione *ad* *hoc*, incaricata di tenere i rapporti con l'OLP e di cooperare per l'organizzazione delle prime elezioni democratiche. Chi parla era uno dei nove membri di quella delegazione. Avemmo, quindi, modo d'incontrare ripetutamente Arafat, che si mostrò come trasformato da quel progetto; ebbe un cambiamento importante di pelle, di orientamento e anche di ideali. Il vecchio rivoluzionario lasciò il posto allo statista, il quale seppe convincere il Parlamento europeo per primo, ma anche l'Europa tutta, che la storia era veramente cambiata. Quello che impressionò gli osservatori europei, una volta che presero visione e contatto ravvicinato con la realtà di Gaza, dei territori e con la realtà palestinese fu che, accanto ad un problema politico, vi era un'emergenza umanitaria, a torto misconosciuta o non sufficientemente sottolineata. cento delle famiglie di Gaza e dei territori viveva, ma vive tuttora, al di sotto della soglia di povertà. Le 675.000 persone ufficialmente censite nei campi profughi dopo la guerra del 1967 erano accampate da più di trent'anni, almeno i sopravvissuti, ancora nelle stesse baracche e nelle stesse condizioni di allora. Qualcuno, con il passare degli anni, chiaramente si attrezzò per vivere un po' meglio, ma passi avanti verso un recupero a livello umano non furono mai compiuti. Va detto che la burocrazia farraginosa e corrotta delle organizzazioni che avevano il compito di

la contraddizione di molte, forse troppe, antenne satellitari, attraverso le quali il mondo occidentale portava in quella miseria immagini di ricchezza, di vita agiata, che non potevano che acuire sentimenti di odio e di rivalsa verso un mondo che non apparteneva a quella gente. Molte erano le sacche di povertà e di emarginazione, come per esempio per gli ex carcerati (più di 200.000 in quel periodo) e per i disoccupati (oltre il 70 per cento), tra i quali si registrava anche una disoccupazione qualificata (più di 30.000 erano i laureati disoccupati ufficialmente segnalati). Il reddito medio di una famiglia palestinese è di circa 300 dollari al mese;

uomini, giovani, donne e soprattutto per far leva sui sentimenti di rivalsa di cui ho parlato prima. Anche l'agricoltura, alla quale si è tentato di dare un impulso con molti fondi europei non ha saputo rispondere all'appello. Hamas, con un'azione molto sapiente (a volte potrebbe apparire perfino subdola), è riuscita a conquistare, ancora nei primi anni, appoggi e simpatie con una presenza nel sociale, con aiuti di carattere umanitario, che altro non era che un modo ripeto, subdolo - per creare forme di arruolamento indiretto. Inoltre, un problema causato dall'inasprimento della lotta armata e da ogni che porta a una recrudescenza nei rapporti tra Israele e la Palestina è quello dei lavoratori migranti, dei pendolari: erano 87.000 nel 1987, oggi pare siano meno di 5.000. Questo perché, ogni volta che si crea o si rinnova un focolaio di tensione, si chiudono le frontiere, quindi vi è gente che perde il posto di lavoro e studenti che non riescono ad andare alla lezioni universitarie. Si era calcolato allora che una giornata di blocco dei lavoratori palestinesi verso Gerusalemme costava

credette veramente fino in fondo nel suo ruolo, non di mediazione, ma di propulsione: mandò in Palestina 600 persone, pagate per organizzare

che da allora ad oggi una serie di eventi catastrofici (dall'11 settembre in poi, al Libano, alla recrudescenza delle vicende all'interno dei Territori) hanno fiaccato indubbiamente questo elemento di speranza e questo momento di possibile recupero della speranza. È per questo che ho voluto ricordare. Se era possibile allora, dopo gli anni terribili dell'origine della crisi palestinese, perché non è possibile recuperare oggi ed aggrapparci a questa possibilità? È questa l'esortazione che vorrei rivolgere al Governo italiano, di farsi promotore anche in Europa di un nuovo slancio, di una nuova linfa di speranza, perché tutti sappiamo che l'Italia è sempre stata *leader* in questa spinta verso la Palestina, commettendo un solo errore.

anche umanitario, vi sia sempre stata sempre una coda politica che ha falsato la nostra immagine ed il nostro ruolo, considerando quella palestinese una vicenda di sinistra, mentre - come ho tentato di dimostrare - è una vicenda che appartiene a tutti nel più profondo della nostra convinzione e nella nostra voglia di esserci per riaccendere, signor Vice Ministro, quella fiamma di speranza.

Il momento forse più produttivo fu quando l'Unione Europea assunse la sua iniziativa per parlare di dialogo: una novità assoluta quella di far parlare gli israeliani e i palestinesi. Ci volle un po' di tempo per far accettare agli israeliani la tesi del dialogo. Gli sviluppi successivi è inutile

certamente l'iniziativa di avere in Libano una presenza militare come pronto soccorso può essere utile, ma non è la soluzione. La soluzione è quella di una

quella che sembrava la guerra tra Libano e Israele, ma che non era la guerra tra Libano e Israele, bensì il constatare che, purtroppo, la questione palestinese è una questione irrisolta. Poi ci sono anche i provocatori: l'iraniano che getta olio sul fuoco con le sue affermazioni straordinarie, per cui certe volte ho l'impressione che sia addirittura una quinta colonna per quanto è stolto nella nella progettazione di determinati indirizzi. In concreto, cosa possiamo fare? Potremmo cercare di sollecitare di nuovo un intervento da parte dell'Unione Europea, tenendo conto che

sensazione effettiva che l'opinione internazionale avverte le loro necessità; in secondo luogo, poiché uno dei punti più dolorosi è la concentrazione, in uno stato assolutamente tristissimo, di oltre mezzo milione di palestinesi in Libano, che il Libano non riconosce, bisogna tentare, magari con un piano di aiuti al Libano, di fare qualcosa per instaurare

frutto di una non sufficiente attenzione a tutto il male che è stato fatto lungo la storia, anche in tempi non lontanissimi, contro il popolo di Israele. Dobbiamo cercare, però, di aiutare a far riflettere. Vi sono stati momenti di speranza quando è stato deciso lo sgombero dei coloni ebrei dalla Striscia di Gaza.

Invece, se si continua a tirare su il muro (signori, noi viviamo in una città in cui si sa bene cosa voleva dire il muro: il muro è il ghetto),

però, io credo che tra gli obiettivi politici che devono essere ripresi dall'Unione Europea questo deve essere un obiettivo prioritario. Ci commuoviamo giustamente quando accadono fatti gravi, come quello dei giorni scorsi, però, fino a che lasceremo che possano contrapporsi, da un lato, una aviazione fortissima, dall'altro dei *kamikaze*, è inutile poi piangere

Ricordiamo quante decisioni sono state prese che davano soddisfazione anche ai palestinesi, ma quando mai sono state poi applicate? Saremo migliori da adesso in poi ? Non lo so. Una cosa sola non deve essere ammessa: la rassegnazione dinanzi ad una situazione che da sola certamente non si correggerà.

Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il Governo per la pronta risposta alla sollecitazione venuta dall'Assemblea del Senato e, in particolare, il vice ministro Intini per la chiarezza, vorrei dire non non solo la lucidità ma anche l'onestà, con la quale ha analizzato la situazione, innanzitutto nei suoi risvolti umani, che sono veramente drammatici. Abbiamo tutti nella mente, negli occhi l'orrore di quelle immagini terribili venute ieri dalla Striscia di Gaza. Insieme al dolore per le vittime, c'è anche lo sdegno per un'ennesima picconata che è stata data, al di là del fatto che è stato denunciato un incidente, alle prospettive della pace. Quel bombardamento terribile ed atroce non solo ha mietuto delle vittime innocenti, in particolare donne e bambini, ma ha riportato indietro le lancette dell'orologio in una situazione critica, sotto il profilo politico. Non mi dilungo perché condivido quanto è stato detto dal vice ministro Intini. Mi soffermo solo su un punto che ha toccato e che credo sia utile sottolineare:

presente in maniera massiccia in quel contesto, al confine tra Israele e Libano. Come ha detto giustamente l'onorevole Intini, abbiamo contribuito in modo - credo - determinante a spegnere un incendio e siamo lì per consentire il mantenimento di una fragilissima tregua che ha un solo possibile significato,

attore, gli Stati Uniti d'America. Le elezioni ci sono state e hanno avuto un risultato chiaro e netto, che ha bocciato una linea di politica estera che, per la verità, già l'Amministrazione in quanto tale aveva riconosciuto, più o meno implicitamente, essere improduttiva e sbagliata con la scelta del nuovo segretario di Stato, Condoleezza Rice. Ora c'è stata la rimozione del segretario alla difesa Rumsfeld. Ebbene, è necessario, come ha detto il Vice ministro, che il Congresso degli Stati Uniti e la Presidenza, in una gestione per forza di cose *bipartisan*, intraprendano un'iniziativa forte in questa direzione.

immediato con il Presidente per esaminare la situazione in Iraq, che naturalmente per il popolo americano continua ad essere la priorità, non fosse altro per la quantità di truppe esposte ogni giorno ad attacchi e ad

per un verso la Siria e per l'altro l'Iran, che è diventato, nei fatti, un paese decisivo per tutti e tre gli scenari attuali di crisi, quello libanese e, in qualche modo, anche quello palestinese, quello iracheno e quello afgano. Infatti, in tutte tre i contesti - è difficile fare una graduatoria di quale sia più degradato e quale

siamo al 9 novembre e non è successo nulla. Evidentemente non è con la logica degli *ultimatum* che si va da qualche parte. Serve un'iniziativa politico-diplomatica serie che coinvolga e responsabilizzi l'Iran come potenza decisiva decisiva in quell'area, perché questa è l'unica strada attraverso la quale possono andare avanti le ragioni della pace. Credo che, sulla base di quanto detto dal vice ministro Intini, il Governo stia facendo quanto in suo potere per attivarsi in questa direzione. Se è possibile, da parte del Parlamento stimolare ulteriormente un rafforzamento di questo impegno, credo che questo sia il significato

Signor Presidente, signor Vice ministro, senza retorica: 19 morti innocenti, forse di più, e fra questi otto bambini, e altri bambini ancora feriti gravemente, mutilati. L'ultima strage di Gaza pesa come un macigno e deve pesare. Deve pesare sul Governo israeliano e sul suo esercito, che continuano a percorrere la strada insensata di rappresaglie segnate, non come diciamo noi ma come dice Amnesty International, da un profondo disprezzo per la vita dei civili palestinesi. Dal 2 novembre, data di inizio della nuova azione militare israeliana contro i palestinesi, i bambini uccisi sono 50. Dobbiamo ricordare che la popolazione della Striscia di Gaza è composta per il 50 per cento da minorenni e che la loro vita, da sempre, è fatta di terrore, denutrizione, reclusione nelle case, senza acqua e elettricità, bambini che non vanno più a scuola, che non godono di altra protezione che non sia quella dei loro genitori, protezione fragile, spesso impotente e perciò disperata. Certo, tutti condanneranno questa strage e tutti, o quasi tutti, come sempre, deploreranno la linea di condotta di uno Stato che perennemente colloca sotto il titolo dell'autodifesa ogni atrocità commessa. Ma condanne e deplorazioni fin qui non hanno indotto Israele a un mutamento di rotta neppure parziale ed è per questo che questa strage deve pesare anche sull'insieme della comunità internazionale e, in primo luogo, voglio dirlo, sul Governo degli Stati Uniti, che più di chiunque altro incoraggia e ha incoraggiato sin qui il permanere della politica israeliana su questa strada insensata. C'è da chiedersi: fino a quando ancora l'appoggio americano incondizionato ad Israele sarà cieco di fronte agli esiti ormai chiarissimi della propria stessa politica? C'è da chiedersi, mi auguro, se continuerà a essere indifferente alla frustrazione, alla collera, alla disperata e disperante violenza che genera in milioni di arabi che circondano Israele, ai quali ancora brucia quella prima risoluzione dell'ONU - è vero, senatore Andreotti - che indicava la soluzione del problema nella creazione di due Stati, soluzione che ha visto uno solo dei due Stati, quello israeliano, svilupparsi e inserirsi nella comunità internazionale, non già quello arabo‑palestinese. Perché, non c'è dubbio, l'insensatezza di quella politica è più evidente che mai e inizia a provocare vere e proprie sconfitte. La sconfitta del presidente Bush con il corollario delle dimissioni del suo Ministro della guerra, la sconfitta di una linea, la quale, fondata sull'unilateralismo ha affidato unicamente alla forza e, di più, alla prepotenza e alla barbarie di guerre senza fine, senza dopoguerra, il problema del terrorismo e dell'instabilità di varie aree del mondo, a cominciare dal Medio Oriente. Non basteranno le condanne e le deplorazioni per la strage di Gaza, ancor meno avranno efficacia gli appelli alla moderazione rivolti ora ai palestinesi. La strage di Gaza chiede giustizia, prima di tutto; giustizia va resa alle vittime; giustizia in luogo della vendetta, subito. Per questo il Consiglio di sicurezza, convocato d'urgenza, deve giungere a una risoluzione rispetto, questa volta molto fermamente. Il nostro Governo, reso più forte dal prestigio guadagnato grazie alla svolta in direzione di una politica di pace, si è attivato, lo riconosciamo con sincerità e anche con grande adesione, ma deve ancor più attivarsi, perché in quella sede si imbocchi con decisione la nuova strada di pace e si faccia di tutto in questa direzione: l'Italia, l'Europa le Nazioni Unite. Soprattutto si incalzi la comunità internazionale, si faccia pressione perché Israele cessi subito definitivamente i e perché a garantire la sicurezza della popolazione palestinese e di quella israeliana sia una forza di interposizione sotto l'egida dell'ONU, come per il Libano. per il Libano. Anche di fronte al calare delle possibilità, che tuttavia non vanno frustrate, di un nuovo Governo palestinese di unità nazionale, occorre operare per per indurre Israele a riaprire un percorso di pace che porti verso l'obiettivo storico della costruzione dello Stato di Palestina, con capitale Gerusalemme Est. Est. È vero, onorevole Intini, tutto si tiene in Medio Oriente, ma la crisi più grave, madre di tutte le crisi, resta il conflitto di Israele contro la Palestina. La fine di questo conflitto è la maggiore garanzia per l'esistenza e la sicurezza stessa di Israele. La chiave del rapporto di Israele con il mondo arabo,

che uscire dalla spirale di violenza con i palestinesi è la condizione principale per rafforzare la loro sicurezza. Questo, come minimo, dobbiamo alle vittime innocenti di Gaza e ai milioni di innocenti che da troppo tempo da noi non si aspettano più nulla. La nostra rassegnazione acquiescente, dobbiamo saperlo, nelle aree martoriate della Terra genera vendetta e violenza all'infinito. Aprire uno spiraglio di speranza, onorevole Intini,

Signor Presidente, esprimo la mia solidarietà alle vittime, e quindi al popolo palestinese, e il ringraziamento al Governo per la prontezza ad affrontare in quest'Aula una pacata riflessione sul problema tragico che oggi si pone davanti a noi. Come è stato detto da altri colleghi, la semplice condanna rischia di essere un puro moto dello spirito, incapace di determinare effetti politici.

di fronte al risultato elettorale di Hamas, che ha sostanzialmente impedito ad Abu Mazen di formare un Governo di unità nazionale, che fosse che fosse un interlocutore serio anche rispetto al Governo di Israele. La guerriglia continua ad attraversare le vie della Palestina e bisogna prendere atto che la pace si fa in due.

accanto e alla base della spirale dell'odio, quella delle provocazioni. È vero che il conflitto tra Israele e Palestina è il punto cruciale del Medio Oriente, però è anche vero che esso è la ragione di strumentalizzazione da parte di altri. Non basta una semplice invocazione di pace. Quando si invoca - correttamente, sotto il profilo dell'analisi politica a cerchi concentrici che arrivano a Damasco e a Teheran, bisogna anche prendere atto dei progetti politici, quelli aperti e quelli non conosciuti, non chiari e non pubblici, che questi due Paesi, questi due Governi, in un rapporto anche contraddittorio tra di loro, tentano di portare avanti. Ci troviamo allora in presenza di un problema che non si risolve con un atteggiamento di pura solidarietà ai palestinesi, ignorando le ragioni della sicurezza di Israele. Chi vuole la pace deve partire da questo punto fermo; la sicurezza di Israele è la condizione perché si faccia la pace, la sicurezza di Israele è la condizione per la quale si faccia lo Stato palestinese. Certo, se andiamo a riguardare la storia lontana (tra il 1945 e il 1948 il mondo occidentale, i vincitori, ma non soltanto i vincitori del mondo occidentale, fecero degli errori gravissimi e quelli in Medio Oriente pesano moltissimo) e torniamo indietro alle origini, non facciamo un passo in avanti; noi abbiamo l'oggi da affrontare.

Il Governo italiano si deve muovere nel quadro del più stretto collegamento, innanzitutto con l'Unione Europea e poi - con molta franchezza - se vogliamo una svolta autentica da parte di Israele, accanto al problema centrale della sua sicurezza, dobbiamo risolvere il problema della fiducia del Governo agli Stati Uniti. Ciò con molto realismo, altrimenti la questione palestinese rischia di far incendiare tutto il Medio Oriente. L'Italia è andata in Libano, ma il timore - ripeto questa espressione che si apra un incendio che va dalla Palestina, da Gaza al Libano, all'Iraq - perché sono, questi sì, anelli di una stessa catena - è molto fondato e va affrontato con realismo politico, con chiarezza di idee, senza abbandoni a preferenze particolari. Se l'Italia vuole assumere un'iniziativa che sia anche di mediazione, tanto difficile, soprattutto perchè nel mondo palestinese c'è ancora da risolvere il problema politico del rapporto tra Abu Mazen e Hamas,

ha assunto sulle sue spalle una responsabilità molto grande in Libano; preghiamo il Signore che tutto possa continuare ad andare bene, ma questo non ci autorizza a fare altri balzi, questo ci autorizza invece a perseverare sulla linea del servizio che si vuole rendere in Libano con coerenza, adesso contribuendo a risolvere il problema palestinese. Ma, ripeto, questo problema si risolve su una linea di confronto, che sarà anche duro e severo, ma non deve rinunciare alla franchezza. La solidarietà ad Israele non può essere mai remissività, soprattutto dinanzi ai rischi della deriva che l'eccesso di paura e di preoccupazione può anche indurre. Sotto questo profilo auspico un'iniziativa politica del Governo, costante e continua, sulla quale il Parlamento penso che abbia il dovere di vigilare e di interloquire efficacemente. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martone.

non fa altro che riempirci di sdegno e di grande preoccupazione per il futuro e le sorti della pace di tutta quella Regione. Vorrei, però, ricordare che l'offensiva israeliana a Gaza va avanti da molto tempo sono ancora vive nella nostra mente le immagini di un altro drammatico episodio, la sparatoria contro un gruppo di donne e ragazze che stavano manifestando, qualche giorno fa. Chi ha visto le immagini è rimasto agghiacciato dalla crudezza e dalla violenza, appunto, che trasmettevano. Questa strage avviene - com'è stato sostenuto anche da parte di altri miei colleghi - in un momento particolarmente delicato, che poteva anche rappresentare l'inizio di una svolta, come giustamente ha anche affermato lei, signor Vice ministro. Hamas e Fatah speriamo che continuino a negoziare la costruzione di un Governo di unità nazionale con tecnici e indipendenti che, appunto, dovrebbero rappresentare il primo segnale di svolta. Leggendo le dichiarazioni dei *leader* di Hamas, sembra che vi sia la volontà politica di compiere un passo in avanti: si parla di Palestina come di un qualcosa di molto più esteso di Fatah e di Hamas e del bene di tutti i Palestinesi come di un qualcosa che deve andare oltre le vecchie separazioni ed i vecchi conflitti. Un Governo di unità nazionale servirà a sbloccare gli aiuti, a cercare di dare un po' di ossigenoall'economia palestinese ormai in ginocchio ed anche - come hanno giustamente ricordato il Vice ministro, ma anche altri miei colleghi - a sbloccare il percorso verso la costruzione di un'iniziativa diplomatica nuova, che abbia maggior vigore e possa certamente costruire le premesse per una Conferenza internazionale di pace per tutto il Medio Oriente. Sono stati centinaia i Palestinesi morti o uccisi dal giugno scorso, quando Israele, appunto, ha scatenato l'offensiva a Gaza, con il pretesto della liberazione del soldato Gilad Shalit. Ieri John Dugard, relatore speciale dell'ONU sui diritti umani, non ha esitato a chiamarla una brutale punizione collettiva contro un popolo. Allora, a queste condizioni, non possiamo rimanere stupiti, pur condannandole,

che ha chiesto la convocazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che appunto si riunisce oggi, perché mi è sembrato un segnale, seppure minimo, ma comunque incoraggiante, del lento processo di trasformazione di Hamas da milizia paramilitare a forza politica, necessariamente avviato dopo la vittoria elettorale, che difatti è lo stesso processo che auspichiamo per Hezbollah, cioè la trasformazione da forza militare o paramilitare in soggetto e attore politico, con tutte quante le conseguenze del caso. Abbiamo poi letto in molti un'offerta di tregua, pubblicata sull'«Herald Tribune» dal consigliere diplomatico di di Haniyeh, che dà la disponibilità ad entrare in una *Hudna* (tregua in arabo) per porre immediatamente fine all'occupazione ed iniziare un periodo di coesistenza pacifica, nel quale ambedue le parti interromperanno ogni provocazione e aggressione militare. Anche questo mi sembra un segnale importante, che non dev'essere lasciato cadere nel vuoto. Altro discorso riguarda Israele: quando discutemmo della ricaduta politica interna, anche culturale, in questo Paese, della disavventura e, comunque sia, della campagna militare in Libano, in molti speravamo che questo portasse un forte ripensamento all'interno dell'*establishment* militare e politico israeliano rispetto alle strategie militari e di sicurezza, e invece così non sembra sia stato. Innanzi tutto, la campagna a Gaza dimostra che quel ritiro unilaterale da Gaza, tanto acclamato da molti, come Ariel Sharon, altro non era se non una continuazione delle occupazioni militari con gli stessi mezzi ma con altri metodi, una sorta di controllo telecomandato dall'esterno. È anche vero, però, che ascoltando le diverse reazioni alla strage da parte di esponenti del Governo israeliano, mi risulta evidente che vi sia ancora una forte discussione interna tra falchi e meno falchi nel Governo, che però continuano a non trovare una sorta di accordo sulla via da seguire: questo va certamente alle spese di un popolo palestinese ormai allo stremo. Siamo preoccupati anche dei recenti sviluppi di politica interna in Israele, con l'ascesa del nuovo vice ministro Liebermann, che certamente ha posizioni che non aiuteranno molto la causa della pace. Vorrei ricordare, per cercare di capire la filosofia di fondo che oggi ispira le forze sane della società civile israeliana, quanto ho letto in un bellissimo discorso tenuto da David Grossman in memoria dell'undicesimo anniversario della morte di Itzhak Rabin, qualche giorno fa. sostiene che questi si era reso conto che la società israeliana non avrebbe potuto sopravvivere a lungo in uno Stato di conflitto irrisolto e che la vita in un clima di terrore, violenza, occupazione e disperazione rappresentava un prezzo che Israele non si poteva permettere di pagare, e ciò vale anche oggi. Io penso che proprio da questa consapevolezza diffusa diffusa nella società civile israeliana, che anche oggi ad Haifa e Tel Aviv manifesta contro questa ultima strage, possa partire la ragione di una costruzione di un negoziato e di una pace duratura ed equa per tutti. I contorni di questa soluzione li ha prospettati di recente anche *l'International* *Crisis* *Group* in un'interessantissima iniziativa sottoscritta da decine e decine di ex Primi ministri e Ministri degli esteri di tutto il mondo. Anche in essa si fa riferimento all'unico possibile punto di ricaduta ricaduta già discusso altre volte anche qui in Parlamento, cioè alla Conferenza internazionale di pace. Oggi, però, dobbiamo capire quali sono i passaggi per arrivare i passaggi per arrivare ad una conferenza che possa finalmente dare pace a quella tormentata regione. Anzitutto, l'Italia e Europa dovranno adoperarsi per raggiungere un «cessate il fuoco». Dovrà seguire l'avvio di colloqui tra la*leadership* palestinese e Israele, possibilmente con la mediazione del quartetto, il supporto della Lega Araba, e anche di altri Paesi chiave, Iran e Siria *in primis*.

Sappiamo che è entrato in vigore ed è stato ratificato da ambedue le parti. Vi chiediamo perlomeno di analizzarlo e verificarne la compatibilità rispetto agli sforzi di pace che cercate di fare. *L'International* *Crisis* *Group* sottolinea che un elemento di discontinuità rispetto ai processi, sempre avviati e mai conclusi, di pacificazione è rappresentato dal protagonismo di un Paese terzo, quello definito mediatore onesto, in inglese «*honest* *broker*». L'Italia potrebbe svolgere con l'Europa questo ruolo anche grazie alla credibilità acquisita nella gestione della difficile crisi libanese e anche nella ricerca estenuante e convinta di una soluzione multilaterale facente perno sulla legalità internazionale. Io sono d'accordo con quanto detto: non possiamo assolutamente abituarci alla rassegnazione né soltanto fermarci a questa ultima strage, la punta di un *iceberg* che sta caratterizzando fin troppo la vita quotidiana di donne, uomini e bambini palestinesi che molte volte incontriamo anche

ma perché la popolazione, e quindi coloro che abitano la zona, hanno avvertito i due esponenti politici. Su questo fatto dell'invio dei missili Qassam la dichiarazione di uno degli abitanti «Loro giocano coi missili e noi moriamo»

Questa è una concezione di normalità che noi rifiutiamo. Credo che la rappresaglia di Israele, forse in questo caso al di fuori di ogni logica, esasperata, provocatoria, venga anche non dico giustificata, ma in parte compresa se consideriamo che ogni giorno da tempo i missili Qassam partono dalla Striscia di Gaza.

visto che ci sono il partito del presidente Sharon e quello socialista e che il ministro della difesa israeliano sia Peretz, cioè un grande esponente del partito socialista.

che esiste in Israele una realtà nuova che, peraltro, è stata verificata non più tardi di qualche mese fa da elezioni certamente libere e democratiche, che sono avvenute in quel Paese. Pertanto, cercare sempre una realtà israeliana che non esiste credo sia un altro tragico errore che si compie nel valutare questa situazione. Aggiungerei un'ulteriore osservazione che non ho sentito. Gaza

cioè che non è stato concordato con la parte palestinese. Anche questo è formalmente vero, tuttavia è formalmente vero che di colloqui tra le autorità israeliane e quelle palestinesi durante il ritiro da Gaza ne sono avvenuti in grande quantità; vorrei ricordare ad esempio l'intervento dell'ex direttore generale della Banca mondiale che sembrava dovesse assumere la veste di garante dal punto di vista economico della trasformazione di Gaza. Ebbene, quella città, che tutti noi ci aspettavamo dovesse diventare l'esempio, l'embrione di un'area autonoma e governata dai palestinesi, in questo periodo ha solo dimostrato la capacità dei palestinesi di proliferare servizi di sicurezza, un inizio di guerra civile che tanto ha preoccupato la stessa Autorità nazionale palestinese. Si tratta, quindi, di una situazione che certamente non depone a favore dell'assunzione di responsabilità e della capacità in questo senso dei palestinesi. Ma questa è solo cronaca.

Voi non parlate più della smilitarizzazione di Hezbollah, non lo facciamo più nemmeno noi; non starò qui a ripetere una polemica nella quale non ho mai creduto. Lei ha detto una cosa ancora più vera quando ha affermato che abbiamo pochissimo tempo, perché abbiamo una finestra di opportunità politica che forse può durare fino alla fine del 2007, tanto per darci un tempo misurato.

un braccio di ferro politico all'interno della realtà libanese perché Hezbollah chiede un Governo di unità nazionale, che è cosa ben diversa dal governo Siniora; cioè di far entrare all'interno della maggioranza il Gruppo di Michel Aoun, che conta 21 deputati su 120 e che certamente risponde agli interessi della Francia che lo ha ospitato in esilio per molti anni e lo ha rinviato,

che, forte della legittimazione avuta da queste vicende ma anche dal voto popolare e dal sapere chiaramente che se saltasse il tappo dell'imbroglio del censimento del 1938,

C'è poi l'altro pilastro, sul quale abbiamo convenuto, del rafforzamento dell'Autorità nazionale palestinese attraverso un Governo di unità nazionale che avrebbe consentito in maniera indiretta anche ad Hamas

da tutto il mondo arabo per fare esplodere le proprie contraddizioni. I palestinesi pagano la drammaticità di un mondo arabo che scatena in Palestina tutte le sue tensioni e contraddizioni nei confronti del mondo occidentale e soprattutto nei confronti del Governo degli Stati Uniti. La vera grande iniziativa su cui siamo disposti a ragionare è come coinvolgere

Lasinistra estrema ha parlato di crimine contro l'umanità. Vorrei ricordare che crimine contro l'umanità è stata la *Shoah*; tutto il resto, quando si tratta di azioni di guerra, rientra in tragiche e infami azioni di guerra. Lo ribadisco perché altrimenti confondiamo i piani di civiltà su cui ci muoviamo.

Bene ha fatto il senatore Andreotti a dichiarare che purtroppo questa strada la conosciamo: è una strada percorsa, ma che troppo spesso non ha portato da nessuna parte.

arabi in generale e comunque contro Israele. Assisteremo al triste rituale, a cui siamo abituati, di bandiere e fantocci bruciati, gente che grida e va dietro striscioni più o meno agghindata o dipinta.

La Presidenza finlandese si rivolge ad entrambe le parti e sollecita, però, i palestinesi a smettere di lanciare missili sul territorio israeliano.

una nota ufficiale del Governo, afferma: «Gli elementi estremisti di Gaza, che continuano a lanciare missili sul territorio israeliano, portano una loro parte di responsabilità». Solo ieri cinque missili kassam sono stati lanciati verso città israeliane, provocando la reazione della *leadership* di Israele. Nel loro comunicato ufficiale, i russi non dimenticano ‑ come ho sentito qui

è proprio questo l'atteggiamento! Quando viene interpellato, il Primo ministro di Giordania afferma: non ne vogliamo sapere niente, né della Striscia di Gaza, né della Cisgiordania, se la vedano loro, ormai noi ne siamo fuori.

dichiarazioni - che siano lasciati soli, perché in questo momento, è vero, sono soli. La realtà è che sono soli. Noi facciamo i «bla, bla, bla», ma loro sono soli.

Basta. A questo punto ci siamo spaventati di fronte a questo nuovo estremismo dell'Iran, mentre vedo che il presidente Bush, dando le nuove responsabilità a Gates, che è palesemente - lo ha dichiarato - alla ricerca di nuovi contatti con l'Iran e con la Siria,

che in Israele si è creato un vuoto, che la gente si è alienata rispetto alla propria identità, non ricorda più chi è, e soprattutto dove la stanno conducendo i suoi governanti. Inoltre, egli afferma che c'è una tale disperazione e che, quando c'è disperazione, c'è distacco dalla nostra stessa identità dai dai nostri valori, dai nostri ricordi. Vorrei che si pensasse un pochino a questo. Ho nel cuore l'immagine palestinese. Sono stata personalmente in Palestina ed ho organizzato, insieme al patriarca latino di Gerusalemme, Sabbah, delle operazioni di conforto ai bambini della Palestina, che non sono curati, altri si trovano in ospedaletti, mentre il più grande ospedale pediatrico è a

Benissimo, è stato citato il bellissimo discorso - invito tutti i colleghi a leggerlo - pronunciato proprio da David Grossman in occasione del ricordo della morte di Rabin. sottolineare la fine di questo discorso perché forse qui ci incontriamo, forse qui possiamo trovare, maggioranza e opposizione, una linea che in politica estera dovrebbe sempre essere quella della civiltà e dell'unità. dell'unità. È vero, democratici e repubblicani in America possono cambiare, ma in politica estera finiscono per fare azioni che si integrano fra di loro, perché hanno questa capacità

parli con loro scavalcando Hamas, parli ai moderati tra loro, coloro che come me e lei si oppongono ad Hamas, al suo modo di agire. Certamente i palestinesi hanno parte della colpa, se ci troviamo in un vicolo cieco. Ma provi a guardare alla maggioranza di questo povero popolo miserabile il cui destino è intrecciato al nostro, La maggior parte di noi comprende che la terra della Palestina e di Israele sarà una terra divisa, che ci sarà uno Stato di Israele. Perciò fermatevi un momento tutti a pensare, guardate all'orlo dell'abisso, pensate quanto siamo vicini a perdere noi quello che abbiamo creato fin qui. Non siamo un popolo da cento anni di guerra, dobbiamo essere anche un popolo di speranza». Credo che il nostro Governo e la nostra azione debbano essere tutti protesi verso questo filo. Non si tratta tanto di questa o quella forza di interposizione, che sappiamo che può lasciare il tempo che trova. L'importante è riuscire a parlare ai popoli, direttamente ai popoli. Scavalchiamo i dirigenti dei popoli che - come giustamente dice Grossman - sono più estremisti delle loro popolazioni, per una sorta di *captatio* *consensi*. Allora, facciamo quest'azione. Benissimo quello che è stato detto sul piano di pace Marshall da parte di Rosenberg qui a Pavia, ma ricordiamo che questo piano fu proposto proprio dal presidente Berlusconi nella precedente legislatura e si fecero tanti sorrisetti sulla richiesta di un piano Marshall e di un momento di unione che stabilisse come intervenire perché i palestinesi potessero avere il loro Stato e gli israeliani potessero avere la loro pace insieme con il loro riconoscimento di popolo e di Stato.

a partire dall'eccidio grave che io condanno, e che quest'Assemblea condanna, ci porta ad essere molto preoccupati per ciò che sta avvenendo. Ha ragione Grossman - come ricordava la senatrice Burani Procaccini

Essere per Israele Paese di speranza vuol dire probabilmente cambiare molto della sua politica; certamente tutti noi riconosciamo i problemi che ci sono, lo ha detto il vice ministro Intini, come sono avvenuti i fatti, ciò che viene dalla Striscia di Gaza ma anche ciò che viene da parte della politica di Israele. La nostra preoccupazione si accompagna all'angoscia che, se non si ferma la spirale della violenza, com'era in Libano quest'estate, potrebbe non esserci una via di ritorno. Forse rispetto al passato questa è la novità politica e storica:

E non giova a nessuno, in primo luogo a Israele. Tutti noi teniamo alla sicurezza di Israele ma anche alla sicurezza degli altri. L'uccisione di bambini, di innocenti, può solo provocare nuovi incendi, allargare un giacimento d'odio molto grave. Qualcuno ha parlato di crimini contro l'umanità; il centro Btselem, il centro israeliano per i diritti umani, ha scritto queste cose ieri, quindi non qualche estremista di sinistra italiano. Le circostanze in cui i palestinesi sono stati uccisi, incluso il fatto che il bombardamento di artiglieria non è stato un'azione difensiva, giustifica il grave timore che l'azione sia un crimine di guerra,

Quindi, c'è qualcosa di più se Grossman dice questo e se il centro di Btselem, parla di ciò. Bisogna evitare di arrivare oltre il confine, oltre cui non si può tornare indietro. La Rice ha espresso ad Abu Mazen una profonda tristezza per la strage; io spero - dirò poi alcune cose in proposito - che l'amministrazione americana vada al di là della costernazione, di cui c'è bisogno ma che non è sufficiente. Questa violenza che colpisce in modo indiscriminato è sicuramente il metodo più sicuro per non ottenere la pace e sta provocando anche una profonda reazione a livello internazionale. Il bilancio dei morti di queste settimane

bisogna fermare le azioni di eccidio, bisogna fermare i razzi Qassam. Beit Hanun deve divenire un momento importante dal punto di vista politico. Dal punto di vista più complessivamente politico, queste azioni e questi eccidi forse puntavano a rinviare, se non a sabotare, la costituzione del Governo di unità nazionale (ha detto Intini che da quelle parti si fa dietrologia, e forse non solo da quelle parti), quel Governo di unità nazionale a cui Abu Mazen ha lavorato insieme ad Hamas. D'altronde, diceva il collega Tonini che questo Governo di unità nazionale è una delle condizioni *sine qua non* per poter avviare una nuova fase.

c'è stata un'idea più che altro di destabilizzazione della Palestina che di trovare un equilibrio positivo con quel territorio. E questa idea forse di destabilizzazione delle forze politiche palestinesi ha portato solo a delegittimare le forze moderate (come dicono alcuni studi, tra l'altro precisi, non solo italiani ma anche americani), ha favorito Hamas e penso che questo elemento di delegittimazione delle forze moderate abbia creato e non possa creare che situazioni negative. Forse sarebbe bene che Israele comprendesse che questo incrudimento della situazione non giova alla sua sicurezza, a cui tutti teniamo, ed è una politica sbagliata che può portare solo in un vicolo cieco. Occorre che ci sì fermi prima che sia troppo tardi. C'è una necessità oggettiva della politica del dialogo; queste non sono petizioni di principio, non c'è alternativa alla via negoziale.

qualche ora fa alla Camera - in primo luogo attraverso il contributo del Governo italiano. In questi mesi le speranze di pace da quel lato sono diventate concrete, ma ricordava giustamente il vice ministro Intini, se non c'è oggi un consolidamento della pace da questa parte,

non penso che sia una cosa qualunque, una forza di interposizione, ma una cosa concreta, seria. Dice giustamente il ministro D'Alema che ci sono delle difficoltà: il contingente può solo essere dispiegato se c'è un accordo delle parti.

le altre forze, l'ONU, la stessa amministrazione americana. Dobbiamo lavorare perché questo avvenga perché sia ad Est sia ad Ovest ci sia una sicurezza tale che permetta di non ampliare l'incendio Questo vuol dire, in primo luogo, lavorare con molta lena, affrontare questo passaggio con una forte concertazione internazionale, come abbiamo fatto nella crisi libanese ripeto - con l'intesa dell'Europa, con gli americani e valorizzando al massimo l'ONU a partire dalla riunione di oggi. Il voto in America e le dimissioni di Rumsfeld,

A partire da ciò, il mio auspicio - ma penso debba essere qualcosa di più - è che la stessa amministrazione americana voglia esercitare la sua influenza su Israele per trovare una via di pace. Non so - come diceva il senatore Mantica - se cambierà.

una soluzione per tutti e aprire il confronto a livello più complessivo del Medio Oriente, affrontando i rapporti con la Siria e con l'Iran. Tutti noi, quando parliamo di questo, non parliamo solo di piccola politica, ma anche di grandi elementi. Voglio concludere con le parole di Carlo Maria Martini: «Non ci sarà pace nel mondo finché non regnerà in quelle terre piena pace. E tutti gli sforzi di pace in quelle terre avranno una ripercussione straordinaria sul pianeta intero».

e non, come riferito all'interrogante, tra il 3 e il 9 luglio - dal comandante di reparto della casa circondariale di Cuneo a personale di polizia penitenziaria che aveva da poco terminato il turno di servizio notturno, e con riferimento ancora alla successiva attivazione di procedimenti, disciplinari prima, penali poi, nei confronti di quanti si erano rifiutati di rendere tale prestazione, si rappresenta quanto segue. I procedimenti disciplinari a carico degli agenti sono stati archiviati dal direttore dell'istituto in data 19 giugno 2006, in considerazione del divieto di utilizzo per più di sei ore del personale che svolge servizio notturno, ai sensi dell'articolo 9, lettera *b*) dell'accordo quadro nazionale vigente. Pendente la successiva denuncia davanti all'autorità giudiziaria degli agenti da parte del comandante di reparto per supposta violazione dell'articolo 329 del codice penale («Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di forza pubblica»), in data 27 giugno 2006, il provveditore regionale competente, ai sensi dell'articolo 31 del decreto ha sollecitato il direttore dell'istituto a sottoporre a procedimento disciplinare il comandante di reparto e a segnalare l'operato dello stesso all'autorità giudiziaria, ravvisando gli estremi di reato previsti dall'articolo 323 del codice penale («Abuso d'ufficio»). Ciò detto, cogliendo lo spirito delle preoccupazioni che hanno mosso l'interrogante, si ritiene che nel caso in esame l'operato del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria non possa in alcun modo essere biasimato.

si rappresenta che, riguardo alla mancata corresponsione al personale di polizia penitenziaria dei buoni pasto, il Dipartimento della giustizia minorile ha assicurato al Ministero della giustizia che si procederà al risanamento delle quote non appena le stesse si renderanno disponibili sull'apposito capitolo di bilancio. Si evidenzia, peraltro, che nel 2005 le organizzazioni sindacali richiesero che al personale venissero corrisposti i buoni pasto in assenza della mensa obbligatoria di servizio, che è stata istituita con decreto registrato all'ufficio del bilancio in data 11 agosto 2006. Per quanto riguarda il quesito relativo alla mancanza di convocazioni delle organizzazioni sindacali da parte dei responsabili dei servizi dell'Amministrazione, il Dipartimento della giustizia minorile rappresenta che presso l'Istituto penale per i minori di Torino si è tenuto un incontro con organizzazioni sindacali in data 30 maggio, cui ne è seguito un altro il 19 ottobre scorso, avente ad oggetto: i criteri per l'indizione di interpello per addetto all'ufficio matricola dell'Istituto penale minorenni di Torino; l'organizzazione dei servizi di polizia penitenziaria presso lo stesso Istituto. All'esito dello stesso, l'Amministrazione ha ribadito la necessità di indire al più presto un interpello per la copertura del posto di servizio di addetto matricola, riservandosi di verificare i requisiti di necessità e urgenza per l'indizione dello stesso. In merito al secondo punto all'ordine del giorno della riunione con le organizzazioni sindacali, l'Amministrazione si è impegnata a convocarle per l'inizio del prossimo anno, al fine di confrontarsi sui criteri di assegnazione dello straordinario, in linea con quanto previsto dall'accordo quadro nazionale e dalla circolare attuativa del competente Dipartimento. Inoltre, è stata proposta la formazione di una commissione paritetica, con delega al direttore dell'Istituto penale minorile, finalizzata all'individuazione di un nuovo modello di organizzazione del servizio della polizia penitenziaria ivi destinata, e sulla presentazione di delegata all'attività di cui sopra e sarà formata da componenti delle organizzazioni sindacali e da componenti indicati dall'Amministrazione.

La generale carenza di personale di polizia penitenziaria nella casa circondariale di Torino determina difficoltà nel garantire la copertura dei posti di servizio essenziali al miglior svolgimento dei compiti istituzionali affidati all'istituto e al suo personale. Ciò nonostante, l'Amministrazione penitenziaria esclude che presso la casa circondariale di Torino il personale di polizia penitenziaria espleti doppi turni di servizio. Può accadere che, in casi eccezionali, il personale smontante si trattenga il tempo necessario all'arrivo del personale subentrante nei medesimi posti di servizio: ma queste ma queste occasionali difficoltà attengono alla fisiologia dell'organizzazione del lavoro nelle strutture complesse; tanto più quando esse sono gravate dalle carenze di organico di cui si è detto. Per quanto attiene alla liquidazione delle missioni e al rimborso delle spese sostenute dal personale, risulta che la direzione dell'istituto abbia già provveduto alla relativa corresponsione fino a tutto il 1° aprile 2006, mentre sta predisponendo il pagamento delle spettanze fino all'agosto 2006. In ogni caso, è sempre stata garantita al personale interessato la liquidazione di acconti e anticipi. Circa le difficoltà di approvvigionamento del vestiario, si fa presente che le attività di distribuzione sono state eseguite conformemente alle richieste pervenute, compatibilmente con le disponibilità di materiale in magazzino. Laddove le disponibilità immediate fossero insufficienti, l'Amministrazione penitenziaria ha predisposto una procedura atta a soddisfare nel più breve tempo possibile le richieste, e risulta che nell'aprile scorso il provveditorato vi abbia fatto ricorso per le necessità degli istituti piemontesi.

accogliendo la sollecitazione dell'interrogante, il Ministero della giustizia ha proceduto a verificare le disfunzioni lamentate nella gestione del personale presso la casa circondariale di Biella. L'amministrazione penitenziaria assicura che le istanze del personale vengono regolarmente protocollate, quale che sia il modo di trasmissione; in particolare, le istanze del personale relative a interpelli e concorsi non solo vengono inoltrate con lettera di trasmissione, ma ai diretti interessati viene rilasciato il relativo numero di protocollo. Quanto ai cambi di turno, la direzione dell'Istituto assicura che il personale in servizio ne viene puntualmente informato. Soltanto in due casi, dovuti a mero disguido, non vi è stata tempestiva comunicazione; e di ciò l'Amministrazione - e il Ministero - si rammarica con gli interessati. Infine, per quanto riguarda l'agente alla quale sarebbero stati negati turni di lavoro agevolati e alla quale sarebbero state imposte prestazioni di lavoro straordinario, la Direzione competente riferisce che l'agente in questione gode attualmente di tali turni ed è stata esonerata dal lavoro straordinario. Presidente, ringrazio il sottosegretario Manconi per avere tempestivamente risposto alle nostre sollecitazioni, un complesso di interrogazioni nel quale veniva rappresentato un disagio rispetto alla criticità degli istituti penitenziari del Piemonte, che certamente il recente indulto non ha migliorato, se non dal punto di vista di una pressione demografica che era diventata eccessiva. Le risposte sono in un certo senso burocratiche, anche se dobbiamo dire che alcune decisioni sono state assunte,

(peraltro espresso oralmente, senza ulteriore formalizzazione) di riprendere un nuovo turno dopo solo quattro ore dalla conclusione del precedente, quindi in palese contravvenzione al divieto di impiegare il personale del Corpo nel giorno di smontante. A ciò aveva fatto seguito una denuncia all'autorità giudiziaria. Il responsabile dell'ordine illegittimo, il comandante del reparto,

che si estrinseca nella mancanza di ogni tutela dei diritti personali e contrattuali, ivi compresa la negazione dei buoni pasti dovuti, lascia sostanzialmente inalterate le ragioni del malcontento,

Per quanto riguarda la questione della casa circondariale di Torino, da più di un anno perdura la mancanza del rimborso dovuto per le spese sostenute in missione dal personale di polizia penitenziaria, a detrimento delle condizione minime, quindi imprescindibili, a tutela e salvaguardia del lavoro. Con riferimento alla casa circondariale di Biella, non si è posto riparo alle condizioni di discriminazione che sono state denunciate, aggravate dall'assoluta indifferenza rispetto alle note di sollecitazione del sindacato alla direzione dell'istituto. Sono in realtà casi diversi, che però non esauriscono un complesso di disfunzioni. Va segnalata, ancora, la questione della casa circondariale di Alessandria-San Michele, oggetto di più di un atto di sindacato ispettivo nell'attuale legislatura, il cui provveditore consente di far esercitare ad un direttore di area C2 le funzioni di direzione appartenenti ad area dirigenziale C3, in palese violazione della legge, e lasciando inoperanti ben due dirigenti formalmente e sostanzialmente in grado di assumere quel ruolo. Il disagio è ben più evidente in Piemonte e Valle d'Aosta, comprendendo anche per taluni aspetti, Lombardia e Triveneto, con i casi eclatanti di Brescia e Padova. In tutti questi casi, onorevole Sottosegretario, emerge palesemente l'inerzia, quando non addirittura una controproducente e non giuridicamente accettabile azione dei vertici della struttura penitenziaria, che vanno dalla direzione di singoli istituti fino a dirigenti di livello regionale. Domandiamo, allora, che cosa attenda il Governo - e questo aspetto non c'è stato nella sua risposta - a fare degli accertamenti rigorosi e a porsi realmente il problema, come non sembra stia facendo nella sostanza, sostanza, se non per quei casi che lei ha citato per aspetti assolutamente minimi. Quindi, riteniamo, onorevole Sottosegretario, che la risposta dell'Esecutivo avrebbe dovuto essere quella di operare una verifica rispetto alla direzione regionale dell'Amministrazione penitenziaria, rispetto ad un'area critica, come quella del Piemonte e della Valle d'Aosta, rispetto alla quale non è stato apportato alcun mutamento a livello di dirigenza regionale, né avviata una seria verifica, capace quantomeno di esaminare nello specifico l'azione di chi è responsabile di un andamento generale. Dunque, rispetto alle questioni dette, potremmo anche andare a fare un esame di qual è stato l'effetto dell'indulto, se c'è stato un miglioramento o un peggioramento della situazione. Certamente, dei 24.413 ex detenuti usciti con il provvedimento dell'indulto, già 1.473 sono rientrati per recidiva e di questi addirittura 1.225 in flagranza di reato. reato. Riteniamo che certamente l'indulto ha cercato di dare una soluzione al problema del sovraffollamento delle carceri, però forse non è sufficiente se non vi è la consapevolezza di dover anche per migliorare le condizioni degli istituti penitenziari e soprattutto del personale impegnato in quest'azione. Purtroppo, i segnali che vengono dalla legge finanziaria

che devono essere affrontate sia con misure finanziarie, sia con un atteggiamento più forte. Si tratta di problematiche che non possono essere rinviate, altrimenti quello diventerà l'anello debole della catena e avremo un personale impegnato

sociale*. Signor Presidente, in relazione all'interrogazione presentata dalla senatrice De Petris si rappresenta quanto segue. Con decreto interministeriale in data 7 novembre 2000 del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia, sono stati approvati lo statuto e il regolamento di previdenza e assistenza dell'ENPAF, trasformato con delibera dell'8 giugno del 2000 in fondazione di diritto privato, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994. La privatizzazione ha novato la natura giuridica dell'ente, lasciando, come per tutte le casse trasformate da soggetti giuridici pubblici a privati, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, immutata l'accezione precipua dell'attività di previdenza e assistenza svolta esclusivamente a favore di liberi professionisti iscritti, tenuti obbligatoriamente al versamento dei contributi a quei fini disposti. Ciò è stato evidenziato, proprio per l'ENPAF, dal TAR del Lazio, che ha affermato che oggi l'ente ha natura giuridica di diritto privato, dal momento della sua nuova regolamentazione, intervenuta con l'approvazione dello statuto. Il processo di privatizzazione, per altro, determina che non siano consentiti, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, del già citato decreto legislativo n. 509 del 1994, finanziamenti pubblici diretti o indiretti o altri ausili pubblici di carattere finanziario. A tal proposito, va subito precisato che il patrimonio immobiliare dell'ENPAF non è stato acquistato in virtù di contributi pubblici, ma unicamente grazie alla contribuzione versata dagli iscritti alla cassa. In proposito, si ribadisce che l'ente riceve contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria versata direttamente dagli iscritti, nonché il contributo dello 0,90 per cento previsto all'articolo 5 della legge n. 395 del 1977. Detto contributo è versato dalle ASL all'ente, ma è trattenuto dalle medesime alle farmacie in sede di liquidazione delle prestazioni farmaceutiche rese in regime di Servizio sanitario nazionale.

del 1998), questo non affluisce più all'ente per essere destinato alla gestione generale, ma successivamente riversato ai titolari di farmacia privata. Per questo motivo, l'ENPAF ha approvato uno specifico regolamento attuativo della succitata disposizione convenzionale vigente. La gestione dello 0,15 per cento è separata da quella dell'ente e a decorrere dal 1° gennaio 2001, ha un proprio bilancio autonomo e separato da quello dell'ENPAF. Ciò premesso, va detto che la normativa statale relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali è inapplicabile alla fondazione ENPAF, come a tutti gli enti previdenziali di diritto privato, siano essi privatizzati, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, o privati, ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996. La questione segnalata dal presidente del Comitato inquilini dell'ENPAF è stata oggetto di contenzioso, sia in sede amministrativa sia dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, e, ancora più di recente, definitivamente risolta dalla Corte costituzionale. Il Comitato fonda le proprie doglianze su un'errata interpretazione della portata della normativa vigente in materia di dismissioni immobiliari, del tutto estranea alla fondazione ENPAF e agli altri enti previdenziali di diritto privato.

l'inapplicabilità agli enti previdenziali privatizzati - e, quindi, all'ENPAF ed alle altre casse previdenziali divenute soggetti di diritto privato della normativa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, intesa a suggerire agli enti pubblici previdenziali diverse forme di gestione del patrimonio immobiliare ispirate al criterio del maggior vantaggio economico sulle dismissioni degli immobili degli enti pubblici previdenziali. Su tale normativa, dopo l'interpretazione autentica del legislatore, è intervenuta la Corte costituzionale, che, con l'ordinanza n. 242 del 2006, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sollevata dal tribunale di Roma. Va aggiunto che la finalità del decreto legislativo n. 104 del 1996 era piuttosto quella di imprimere un particolare impulso all'attività di gestione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali, con l'evidente obiettivo di favorire il risanamento della finanza pubblica, che non quello di produrre l'immediata costituzione di un vincolo giuridico in capo all'ente locatore di trasferire la proprietà del bene ai conduttori. Poiché nel momento in cui sono stati definiti con certezza (vedi articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, nella legge n. 410 del 2001) termini e modalità per l'esercizio, da parte dei conduttori, del diritto di prelazione per l'acquisto delle abitazioni, era già avvenuta legittimamente la trasformazione dell'ENPAF in soggetto di diritto privato, appare non in linea con la normativa sopra delineata che tale ente debba essere ancora soggetto alle speciali procedure di vendita delle case previste per il patrimonio immobiliare pubblico, con esiti che risultano palesemente inefficaci per le finanze dello Stato e densi di rischi per l'assetto dell'ente. Gli enti privati sono, infatti, tenuti ad adottare criteri di gestione e piani di investimento prudenziali che tengano conto della contemperazione del rischio degli stessi relativamente alla tenuta degli equilibri di bilancio che devono assicurare, nel lungo periodo, il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali ai loro iscritti, su cui grava l'obbligo della contribuzione. Per questo non si può ritenere che vi sia un obbligo dell'ENPAF alla dismissione o comunque che all'atto della decisione dell'ente di vendere taluni propri immobili la dismissione vada indirizzata esclusivamente ai conduttori. Un eventuale obbligo di vendere il patrimonio immobiliare può rappresentare anzi per gli enti privatizzati un rischio di depauperamento del patrimonio stesso che è invece finalizzato a garantire la liquidazione delle future prestazioni che per gli iscritti risultano essere diritti previdenziali, per loro natura, indisponibili. Il rischio, pertanto, di creare eventuali situazioni di disavanzo di bilancio conseguenti alla vendita del patrimonio immobiliare dell'ente potrebbe esporre altresì le amministrazioni vigilanti a future ed eventuali azioni giudiziarie di risarcimento promosse dagli iscritti dell'ENPAF. Per quanto riguarda i processi di dismissione che hanno interessato il patrimonio immobiliare dell'ENPAF, si evidenzia che gli stessi sono avvenuti attraverso specifici accordi con le organizzazioni sindacali degli inquilini e con la concessione agli inquilini del diritto di prelazione. In particolare, la fondazione, anche a fronte delle aspettative maturate tra gli inquilini che rientravano in programmi di dismissione pubblici, ai sensi della circolare Salvi del 26 agosto 1999, ha concluso, in data 29 settembre 2003, un accordo con le organizzazioni sindacali degli inquilini (SUNIA, SICET e Unione Inquilini) con il quale sono stati definiti pattiziamente criteri e modalità per la vendita agli inquilini medesimi di una parte del patrimonio immobiliare ad uso residenziale. In forza di tale accordo, le procedure di dismissione a Roma Tuscolano e Ostia Lido sono state già al tempo definite con la totalità degli inquilini che hanno acquistato direttamente l'abitazione condotta in locazione. Anche l'alienazione dell'antico fabbricato di proprietà dell'ente a Milano, realizzata nell'anno 2002, è stata disposta previo confronto con le organizzazioni sindacali degli inquilini. Successivamente a tali dismissioni, il 14 ottobre 2004 è intervenuto un nuovo accordo con le organizzazioni sindacali degli inquilini per la cessione in blocco di un ulteriore stabile sito a Roma, in via Rossini n. composto da 44 appartamenti e realizzata l'anno successivo con la contestuale fissazione dei criteri e delle modalità di vendita. Il predetto accordo è stato siglato, come i precedenti, in attuazione dell'accordo integrativo nazionale sottoscritto tra l'ente e le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative in data 6 febbraio 2002, ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998. Per di più, in forza del nuovo accordo integrativo nazionale, sottoscritto in data 31 gennaio 2005, sono state pattiziamente stabilite, in data 12 aprile 2006. tra la fondazione ENPAF e le organizzazioni sindacali degli inquilini SUNIA, SICET, Unione Inquilini e FEDERCASA, le modalità di cessione in blocco agli inquilini organizzati in cooperative del restante patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente ubicato in Ostia Lido. Con l'accordo, oltre 400 famiglie entro il corrente mese diverranno proprietarie delle unità abitative condotte in locazione, mentre per coloro che non sono nella possibilità di farlo le cooperative degli inquilini hanno previsto specifici meccanismi di tutela. Per quanto concerne il contenzioso, richiamato nella interrogazione, instaurato in particolare dagli inquilini degli immobili di pregio ubicati in Roma Eur non oggetto di programmi di dismissione, si osserva che se è vero che la Corte dei conti ha rilevato, nella relazione riguardante il periodo 1999‑2002, l'aumento degli oneri per le spese legali che l'ente ha sostenuto per difendersi dalle pretese avverse, nel contempo ha riscontrato che, se quelle pretese fossero andate a buon fine, l'esito sfavorevole del contenzioso si sarebbe sicuramente riflesso, almeno nel breve periodo, sulla composizione dell'attivo patrimoniale della fondazione del quale gli immobili rappresentavano, e tuttora rappresentano, una componente di peso. In sostanza, pur con la raccomandazione di diminuire gli oneri per spese legali, la Corte dei conti ha rilevato la necessità di quelle spese per tutelare il patrimonio immobiliare dell'ENPAF. L'ente ha comunque tenuto a precisare che le spese legali per la difesa del patrimonio immobiliare, comprensive anche delle azioni per morosità, i cui importi sono oggetto di recupero da parte dell'ente, sono state, nel 2002, pari a 242.998,31 euro. Tali spese sono progressivamente diminuite nel corso degli esercizi successivi al 2002. Analoga considerazione è stata esposta dalla Corte dei conti, sezione controllo enti, nell'ultima relazione al Parlamento relativa agli esercizi 2003-2004. In merito all'ordine del giorno approvato il 23 luglio 2004, l'ENPAF è tra le poche casse privatizzate che hanno stipulato sin dal 2002 con le organizzazioni sindacali degli inquilini un accordo integrativo nazionale e un accordo integrativo territoriale per l'area metropolitana di Roma allo scopo di stabilire: il primo le condizioni normative e il secondo quelle economiche per il rinnovo dei contratti di locazione delle unità ad uso abitativo. In particolare, l'accordo nazionale riconosce agli inquilini il diritto di prelazione nell'ipotesi in cui l'ENPAF optasse per la vendita del proprio patrimonio immobiliare e, comunque, eventuali e futuri programmi di dismissione immobiliare saranno oggetto di specifico confronto con le organizzazioni sindacali degli inquilini. Tali accordi sono stati recentemente rinnovati per il biennio 2005-2006. Si informa, infine, che il 17 ottobre ultimo scorso si è tenuto presso questo Ministero un incontro di carattere ricognitivo in merito all'andamento delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare dell'ENPAF e che nel corso dell'incontro è emerso che il peso delle attività finanziarie immobiliari dell'ENPAF, rispetto all'intera gestione patrimoniale, si è notevolmente ridotto nel tempo. Vista la natura giuridica dell'ENPAF, le amministrazioni vigilanti non possono obbligare l'ente all'alienazione di specifiche unità abitative se l'ente stesso, sulla base di proprie valutazioni gestionali che evidenziano una redditività netta in perdita, non ne stabilisca la cessione. Pur in assenza di obblighi in merito, tutte le operazioni di dismissione, anche quelle realizzate a ente ormai privatizzato, sono avvenute previa la sottoscrizione di accordi con le sigle sindacali rappresentative degli inquilini, allo scopo di concordare specifiche tutele per le fasce deboli, nonché prezzi agevolati di locazione a metro quadro. La questione relativa agli immobili ENPAF appartenenti al blocco Roma EUR non può essere posta a confronto, così come suggerito dal comitato inquilini, con quella che ha coinvolto recentemente l'INPDAP, con riferimento ad immobili situati nella stessa zona metropolitana, in quanto la natura giuridica degli enti, e quindi il quadro normativo di riferimento nei due casi sono diversi. Considerato anche quanto espresso dalle organizzazioni sindacali presenti che rappresentavano gli inquilini, le modalità procedimentali assunte dall'ENPAF, soprattutto nella fase di definizione degli accordi preliminari, sembrerebbero rappresentare una prassi condivisa e, dunque, efficace e positiva sia per i bilanci dell'ente, che per le aspettative degli inquilini.

Rilevo, tra l'altro, una strana e anche un po' impressionante continuità tra la sua risposta a questa interrogazione e risposte precedenti che, peraltro,

mettere in discussione che si possa continuare a ritenere legittima la privatizzazione, perché sia il contributo dello 0,90 per cento che quello dello 0,15 per cento non sono, secondo la risposta del Sottosegretario,

e ripetutamente sui bilanci delle ASL, anche se viene attribuito all'ente attraverso il sistema delle trattenute ai farmacisti. Da questo punto di vista, continuo ad insistere

come un ente non sottoposto alle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare. Quindi, anche riguardo ai presupposti sulla possibilità di essere privatizzato,

i sindacati, si era avviato un processo di conciliazione con gli inquilini. Questi ultimi avevano ricevuto la lettera in cui l'ente manifestava l'intento di dismettere ed avevano, tra l'altro, manifestato